proiettile a Cinzia Bottene, la responsabile del comitato «No Dal Molin». Al di là delle idee che possono essere presenti nel Senato, credo sia giusto che lei le esprima la nostra solidarietà e che si segnalino alle autorità competenti tutti i necessari provvedimenti. Confido, per i buoni rapporti esistenti sul territorio, che già prefettura e questura siano intervenute;

Non si tratta tanto di una questione di Islam o di donne, ma della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà; non è questione di poco conto. Credo che anche nella scelta delle priorità si evidenzino alcune sensibilità.

Senatrice, ricordo benissimo la sua richiesta e la mia risposta; non mi sfugge assolutamente il rilievo della questione che viene posta con la sua richiesta, un rilievo enorme sotto il profilo umano, morale, ma anche economico per il nostro Paese.

di martedì prossimo, decideremo, assieme ai Capigruppo, sulle priorità che ci restano fino al momento della presumibile chiusura. Ovviamente, senza averne discusso con i Capigruppo, non mi posso impegnare a dirle di

prevede che i professori ordinari per poter accedere al CSM non debbano avere alcun altro requisito, mentre gli avvocati devono avere esercitato per almeno quindici anni. L'articolo 135,

servizio. Con questi presupposti, dichiaro il mio voto di astensione, perché non condivido il testo del Governo ma ritengo che anche l'emendamento sia in qualche modo viziato.

in sua assenza, al Sottosegretario per far presente il grave imbarazzo che io personalmente e credo molti altri senatori della Repubblica sentono in questo momento. ho avuto modo di sapere, attraverso le rassegne stampa, che il Ministro avrebbe compiuto un atto: quello di

anche in quest'Aula dal Ministro o dal Sottosegretario), perché non c'era niente di deciso e di determinato e la riforma dell'ordinamento giudiziario poteva cambiare. Signor Presidente,

che sta avvenendo: chieda che venga sospesa questa discussione e che il provvedimento (come avevamo richiesto noi, ma in modo diverso) torni in Commissione. E se la nuova Costituzione materiale va intesa nel senso che in Italia non si possono fare leggi senza che queste vengano trattate con l'Associazione nazionale magistrati io non mi meraviglio, signor Ministro, però non ci chieda di stare qui a votare, a discutere e ad approvare, qualunque sia la proposta che andrà avanti, una riforma dell'ordinamento giudiziario con una dichiarazione impegnativa da parte sua nel senso di «non fate sciopero, perché vi prometto che questa riforma cambierà».

che quando ho fatto riferimento alla possibilità di emendabilità e di miglioramento non mi rivolgevo a chi era fuori da quest'Aula, ma alla mia maggioranza e all'opposizione, nella normale, corretta dialettica parlamentare, pur nel rispetto delle autonomie di poteri e di compiti, e quindi giurisdizioni diverse. Se poi vuole la mia opinione da questo punto di vista, di uno che è un po' indisciplinato, sono dispiaciuto per quanto accade all'esterno, nel senso richiamato ieri, a bagliori di guerra che mi auguro non permangano, che finiscono per appesantire l'atmosfera politica e istituzionale del nostro Paese. Quindi chiedo a tutti di ragionare con molta severità, scevri da pregiudizi ideologici, e di discutere con serenità. La stessa serenità che sto vedendo - e di questo ringrazio le parti in causa - in questo luogo, nella dualità del Parlamento italiano, e spero che l'incamminamento vada soltanto in tale direzione.

mitigando le asprezze, smussando gli angoli, levigando gli spigoli, perché ritengo che questo sia il modo di fare, rivendicando anche a me stesso il primato della politica.

non proseguire proprio nella maniera identica di ieri, chiedo che venga disposta la votazione con sistema elettronico.

si verificano le condizioni per la richiesta del voto elettronico la seduta va sospesa. In questo momento la seduta è sospesa e non capisco come ella stia dando ai colleghi facoltà di intervenire. Se ciò sta avvenendo, che non costituisca precedente, perché la seduta in questo momento è sospesa.

l'emendamento 1.210 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.206.

di comprovare la conoscenza della cultura non solo italiana, ma anche napoletana, sfatando così un mito negativo che da sempre - ahimè - accompagna la Lega.

che creò un certo dispiacere al senatore Manzione quando lui, parlando di me, disse: «Anche il centro-destra ha il suo Manzione». Il senatore Manzione si inquietò ed io rimasi onorato di questa comparazione. Ora vorrei parlare con la serenità anche del relatore. Presidente,veniamo al problema. Secondo il testo di legge varato dalla Commissione il concorso in magistratura, cioè gli scritti, si possono svolgere in più sedi,

in considerazione del fatto che numerosissimi sono i candidati al concorso in magistratura, immaginare più sedi è un modo di rendere più facile l'esecuzione pratica della prova scritta. Benissimo.

è destinato inevitabilmente a ridursi e ulteriormente a contrarsi in relazione agli esiti della prova quiz. La domanda che pongo è allora

il problema era la sorveglianza nel corso delle prove scritte. Non riesco allora davvero a comprendere, non essendovi una necessità di tipo logistico e pratico, perché dovete correre il rischio di consentire che lo svolgimento delle prove scritte, le uniche sicuramente in ordine alle quali non può intervenire alcuna raccomandazione, debbano avvenire in più sedi e quindi con sorveglianze e vigilanze completamente diverse, creando indubitabilmente una disparità di trattamento. senza che nessuno me ne voglia, che anche in questo caso, ove si dovesse abolire la previsione dipiù sedi, non vi sarebbe alcun disastro di natura politica, né vi sarebbe un ulteriore irrigidimento da parte dell'Associazione nazionale magistrati.

che ha ritenuto fosse meglio la sede unica. Personalmente continuo a pensare che invece sia meglio perseguire la via della diffusione nel Paese di queste attività. Certo, c'è il problema che il senatore Palma ha denunciato e io stesso ho evidenziato

cercando di superare le stranezze di questo Paese, per le quali viene considerato normale, ad esempio, in alcuni concorsi di fondamentale importanza, mantenere un certo lassismo.

essere) un concorso per l'accesso alla magistratura a Milano: sarebbe una novità simbolica, però anche molto significativa. Inoltre ho segnalato ieri che, che, anche tenendosi un unico concorso in quel di Roma, vengono fuori dei risultati che, quantomeno dal punto di vista statistico, sono curiosi e sarebbero meritevoli di un qualche approfondimento. Dunque,

credo, molto esperti di esami e di concorsi e sappiamo che quando si è in pochi si lavora meglio, sia da parte degli esaminandi che da parte degli esaminatori. In secondo luogo, mi pare che vi sia un significato simbolico che, almeno

questo emendamento è abbastanza corposo ma in realtà comporta una differenza minima rispetto al testo del disegno di legge in esame. Sostanzialmente propone che la durata del fuori ruolo dei magistrati impegnati nel comitato di controllo sia prevista per la durata dell'attività del comitato e non per la durata dalla prova, perché, essendo una novità questa del comitato che svolgerà le sue funzioni in altra sede, come facciamo ad essere sicuri che non ci sia una qualche coda di qualsiasi natura per la sua attività? Finite le prove, invece, il magistrato deve tornare ad esercitare la giurisdizione. È chiaro che, se ci fosse bisogno di qualche attività postuma, non potrebbe svolgerla perché è evidente che un magistrato che torna in ruolo non può svolgere altre attività. Credo pertanto che l'emendamento che noi abbiamo proposto sia più conservativo e invece la vostra versione più pericolosa perché pone una misura cogente oltre la quale non si può andare. Si tratta semplicemente di una questione di natura tecnica che pregherei il Governo e il relatore di valutare.

Signor Presidente, questo è uno di quegli emendamenti su cui il parere contrario del relatore e del Governo è assolutamente sorprendente. Il tema in discussione è quello dell'incompatibilità di coloro i quali sono chiamati a svolgere la funzione di commissario d'esame per l'accesso in magistratura con coloro i quali hanno in precedenza svolto attività di docenza - così recita il testo nelle scuole di preparazione agli esami. Credo sia assolutamente intuitiva la buona ragione che ha indotto non ricordo chi dei colleghi a presentare l'emendamento che, approvato dalla Commissione, ha modificato il testo originario del Governo. Le parole chiave di questo comma - che non sto a leggere interamente per non perdere tempo - sono le seguenti: «Non possono essere nominati componenti della Commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario». Ora, mi spiace che siano stati aggiunti anche i professori universitari (se ne risentirà il senatore Valditara): probabilmente a questi l'incompatibilità dovrebbe essere tolta, perché ontologicamente al di sopra di ogni sospetto; ma tant'è. Nell'emendamento che propongo, chiedo che siano operati nella sostanza, sottosegretario Scotti, due interventi: che siano sostituite le dizioni «professori universitari» e «magistrati» e che siano sostituite con una più generica riferita a coloro i quali hanno prestato non attività di docenza - che mi sembra assolutamente limitativo - nelle suddette scuole, ma qualsiasi tipo di attività, anche per esempio di carattere amministrativo, insomma che abbiano preso parte a quel fenomeno scuola. Chiedo inoltre - e questa è la terza questione che ritengo debba essere oggetto di perfezionamento dell'intervento normativo, che peraltro condivido - che sia stabilito che la scuola può essere organizzata in qualsivoglia maniera.

la loro collaborazione alle scuole; in secondo luogo, che la collaborazione sia di qualunque tipo e non limitata alla pura e semplice docenza; in terzo luogo, che si estenda alla scuola, in qualunque maniera essa sia organizzata. Si tratta di un emendamento che non ha alcun carattere ostruzionistico, che credo abbia semplicemente contenuti di perfezionamento di una - ripeto condivisibile disposizione introdotta dalla Commissione. Mi domando per quale ragione sia il Governo sia il relatore abbiano espresso parere contrario, peraltro senza fornire alcuna motivazione, con la conseguenza che la mancanza di motivazione sembra essere una sorta di consenso alla non trasparenza, posto che l'emendamento, al contrario, genera maggiore trasparenza.

Faccio presente che il testo che il senatore Caruso vuole emendare costituisce un emendamento all'originario testo a seguito di una mia proposta emendativa in fase referente. Condivido pienamente le affermazioni del senatore Caruso, del senatore Caruso, perché il suo testo è sicuramente, nell'unicità dell'obiettivo, migliore di quello della Commissione. Vorrei aggiungere solo che ciò

di cui al testo che si vuole emendare, proprio perché quel testo fa riferimento ai magistrati e ai professori universitari e non anche agli avvocati, che invece sono chiamati a far parte della commissione di concorso. In definitiva, poiché sostanzialmente lo scopo che si vuole raggiungere è assolutamente comune e siccome non v'è dubbio che nella sua scrittura più completa, per un verso, e più specifica, per altri versi,

a voler riconsiderare i propri pareri quando, in tutta evidenza, le motivazioni offerte lo meriterebbero. Credo sia cosa assolutamente non dovuta da parte sua, lei che certamente ascolta le motivazioni che tutti noi ci sforziamo di offrire, quando si trova a condividere, come immagino abbia condiviso, quelle motivazioni, forse potrebbe sospingere il silente Ministro a

Mi limito a dire - i collaboratori della Presidenza se ne saranno già avveduti - che il testo non è straordinario dal punto di vista della leggibilità, ma forse le parole: «cinque professori universitari»

approvato, ne guadagnerebbe. Chiedo scusa ai colleghi per avere non volontariamente procurato questo disagio all'Assemblea.

nella sua grandissima capacità di votare con tutte e due le mani e di girare contemporaneamente il giornale. Le chiedo un suo autorevole intervento.

maggiore trasparenza. Invito il collega, testé intervenuto richiamando l'Assemblea a qualcosa di molto simile alla trasparenza, di fare lui un esercizio di voto con riferimento a questo emendamento votando a favore e quindi impedendo che vi possano essere imbarazzanti situazioni di partecipanti ai concorsi per accesso alla magistratura nella veste di commissari d'esame che abbiano fino al giorno prima

vorrei testimoniare che quando le proposte dell'opposizione sono condivisibili è giusto accoglierle. Nella specie, questo emendamento 1.216 del collega Caruso interviene su quella parte dell'articolo 1 che detta le norme per la nomina della commissione prevista per i concorsi in magistratura.

per coloro che abbiano svolto, a qualsiasi titolo e modo, nei dieci anni precedenti attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato onorario. Questa forma di anomala innominabilità per le altre categorie che compongono la commissione, cioè i magistrati e i professori universitari; l'intervento del collega Caruso è molto puntuale perché prevede di integrare la norma con l'altra categoria

un atteggiamento dispotico, dispettoso o preconcetto. Questa maggioranza, in Aula, come in Comitato e in Commissione, ha accolto moltissimi emendamenti dell'opposizione si è trattato di una concessione gentile: è stato il riconoscimento di una partecipazione convinta, competente ed effettiva ad un percorso di costruzione di un testo che, mi fa piacere sentirlo dire anche dal Ministro, è largamente condiviso da tutti. Quindi, possiamo in merito sgombrare il campo: il presepe è bello e quando è bello siamo pronti a riconoscerlo. In questo caso il collega Caruso ha confezionato un ottimo emendamento e siamo felici di poterlo votare.

Ora, se non ho capito male il collega Manzione ha dichiarato che ci troviamo di fronte a un testo largamente condiviso;

Lasciamo perdere la riforma della scorsa legislatura, che porta il mio nome e che va cancellata perché ha il gravissimo peccato originale di essere stata scritta dal Parlamento e non dal CSM e dall'Associazione nazionale magistrati, quindi è uno scandalo e pertanto

è un testo che renderà assolutamente succubi i singoli magistrati e quindi è assolutamente anticostituzionale. Ovviamente questo non ci ha impedito di cercare di migliorare da un punto di vista tecnico ciò che era migliorabile, ma ma ciò non implica in alcun modo un'adesione al testo, che riteniamo assolutamente sbagliato e soprattutto umiliante per il Parlamento.

la verità dei fatti e stiamo legiferando su testi di questa natura. Continuo a dire che ritengo anche umiliante il fatto che né il relatore né, soprattutto, il Governo quando rilasciano, a termini di Regolamento, i pareri sugli emendamenti dell'opposizione si degnano di dare una motivazione.

dell'emendamento 1.218 che si propone - anche in tal caso in chiave non ostruzionistica, ma di semplice proposta di perfezionamento del testo - di introdurre un limite di età massimo indipendentemente dal periodo che è decorso dal momento in cui il componente della Commissione è stato collocato a riposo. La finalità è assolutamente evidente; non vi è alcuna ragione per precludere la possibilità di svolgere la funzione di commissario a colui il quale sia stato collocato a riposo, al pensionato, anzi, mi sembra un'idea pregevole perché recupera risorse anche importanti e di rilievo. Tuttavia introdurre un limite massimo di età mi sembra opportuno, anche per ad un certo livello, ad un certo punto, la forbice di distanza tra l'esaminato e l'esaminando, che diversamente potrebbe diventare incongrua.

qualche emendamento intelligente viene proposto, può essere anche accolto. Mi pareva che questo secondo emendamento fosse più che ragionevole nel senso di porre un tetto a anche per non incorrere nello sfruttamento senile e non più minorile: lasciamo a riposo questi professori universitari che hanno quasi raggiunto la soglia dell'ottantesimo anno di età.

È emerso dal dibattito che c'è stata una grossissima ingerenza dell'Associazione nazionale magistrati; mi pare che del resto il sottosegretario Scotti sia

nel corso dell'*iter* istruttorio in Commissione giustizia. Mi riferisco al collega Casson, che ha affermato che c'è stata la totale chiusura da parte dell'opposizione nel collaborare alla stesura del testo finale. Ma delle due l'una: o c'è stato il grande inciucio e ha ragione Di Pietro - e forse lo metto in dubbio, anzi sicuramente - o ha ragione Casson e Di Pietro è una persona che non dice il vero. Veniamo al punto della situazione: è possibile che lasciamo che l'Associazione nazionale magistrati decida quali sono le leggi buone e quelle che non lo sono? Ma qual è il ruolo dell'Associazione nazionale magistrati e, a questo punto, della magistratura in questo Paese? Applicarle, le leggi, o partecipare al processo formativo giudicando e impedendo, a questo punto, leggi che non sono gradite? Ma il ruolo di quest'Aula qual è? È forse quello di fare sentenze? E se noi non possiamo fare leggi perché chi dovrebbe applicarle ed emettere sentenze si sostituisce a noi, cosa è, una sovversione dell'ordine costituito? Vorrei riproporre Montesquieu a tanti magistrati che si permettono di agire in totale libertà in questo frangente. è imputabile soltanto al Capo dello Stato ed è l'attentato alla Costituzione, è così specifico da non potersi estendere o applicare per analogia, ma l'insubordinazione di un un ordine, di un potere all'interno dello Stato non rischia di invadere la sfera di un reato, appunto, di insubordinazione, di attentato alla Costituzione? Qua si stravolgono addirittura i ruoli. Mi rivolgo al Di Pietro politico adesso, non più Ministro: come fa un esponente politico a dire: «Io sto con i magistrati»? Non ha certo ricevuto i voti dai magistrati, Di Pietro, è un libero eletto con i voti degli italiani e dovrebbe dire: «Io rappresento il popolo italiano» e il popolo italiano ha bisogno di una giustizia fatta per il popolo, non a misura dei magistrati *(Applausi dal

altrettanto abbiamo fatto nel corso della legislatura passata, ma sullo sfondo della trattazione di queste materie aleggia sempre il grande tema fortemente avvertito non soltanto dagli operatori della giustizia, ma anche dall'opinione pubblica: quello della separazione delle carriere. La separazione delle carriere però è un argomento che viene rifiutato, il Parlamento da tempo si tormenta su tutte le ipotesi possibili, ma questo tema è un tema rifiutato, è un tema che comporterebbe fatalmente anche una riforma costituzionale, certamente distante dalle argomentazioni delle quali oggi stiamo discutendo. Però è il problema, il vero problema della condizione magistratuale, questa commistione tra accusa e giudizio rifiutata dalla norma costituzionale e comunque sussistente nonostante le pulsioni culturali contrarie. E allora, l'emendamento non intende assolutamente costituire il prodromo di una riforma che prima o poi certamente si farà ma che io vedo ancora molto lontana. tuttavia sia non inopportuno che un giovane magistrato che si appresta ad affrontare una complessa attività possa rappresentare quali siano le sue attitudini di massima, quale attività intenda prevalentemente svolgere, quella requirente o quella giudicante, senza che ciò possa possa minimamente turbare lo svolgimento della sua attività o le valutazioni che in ordine a questa attività si faranno successivamente. Voglio ricordare che la legge Castelli, che con tanta pervicacia si vuole abrogare, su questo tema stabiliva in termini netti una dichiarazione da parte del soggetto che accedeva alla magistratura. La formula che si adotta in questa sede è molto più cauta, molto più blanda, è una dichiarazione di intenti che certamente potrebbe essere sostanzialmente modificata nelle valutazioni più intime dello stesso candidato nel momento in cui, nel corso della sua attività, si rendesse conto che l'una condizione o l'altra siano più apprezzabili rispetto a quelle ipotizzate all'inizio della carriera. Credo che ciò non cambi nulla nella sostanza, di un elemento che può essere introdotto; potrebbe essere un segnale, signor Presidente, ai 200.000 avvocati che reclamano la separazione delle carriere e che invano attendono un segnale dal Parlamento. Rassegno queste mie riflessioni all'Assemblea, perché le consideri e possa fare delle valutazioni che non siano del tutto distoniche rispetto ad un'area della società non secondaria come l'avvocatura italiana.

l'emendamento aveva l'intenzione, almeno io credo, di consentire l'introduzione di una qualche informazione di natura statistica; perché è del tutto evidente

informazioni poteva servire anche al CSM (anzi, soprattutto a quest'ultimo) per valutare in che modo potessero essere coperti i ruoli vacanti. Ebbene, la cosa fa talmente paura all'Associazione nazionale magistrati e alla magistratura organizzata che non può essere nemmeno evocata: fa venire in mente quelle frasi che compaiono in certi libri di fantascienza di serie B, quando il mostro o il diavolo non può nemmeno essere evocato ma basta l'evocazione del nome perché in qualche modo esso si materializzi.

non si capisce neanche più perché, in quanto nella scorsa legislatura si pensava che in qualche modo potesse avere un qualche vantaggio politico a farlo. Oggi la divulgazione di alcune intercettazioni ha dimostrato che ormai (giustamente, da questo punto di vista) la magistratura è fuori controllo: la sinistra, che forse si illudeva di controllarla, di averla alleata si è dovuta amaramente risvegliare da questo tranquillo sogno. sogno. Stiamo creando un mostro che ci mangerà tutti. Questa, purtroppo, è una profezia da Cassandra ma - vedete - c'è un piccolo problema: Cassandra aveva ragione.

l'altra riforma, quella che portava la firma dell'allora ministro Castelli. Lo voglio ricordare non per fomentare polemiche o climi di contrapposizione, ma soltanto perché c'è una storia che lega le cose e i comportamenti. Se quella storia in qualche modo resta libera nella mia memoria, ritengo necessario intervenire come maggioranza per evitare di commettere quello che all'epoca, secondo me, fu un errore

a discutere approvando anche gli emendamenti che condividiamo, perché è evidente che la maggioranza deve farsi carico di realizzare attraverso i disegni di legge il programma di Governo per il quale è stata eletta.

emendamenti dell'opposizione. Questo è il metodo di una maggioranza responsabile, che è pronta a misurarsi concretamente e non ha bisogno d'imporre in qualche modo i muscoli per cercare di accreditare una convergenza che sia effettivamente condivisa. Questo perché, è innegabile, siamo una maggioranza abbastanza plurale, ecco perché il lavoro proficuo svolto in Commissione ha prodotto il testo condiviso che abbiamo in Aula. Occorre però anche ragionare di quello che significa questo testo rispetto al decreto legislativo n. 160 che è stato modificato. Le novità più rilevanti - ne hanno parlato in pochi fra i colleghi - sono due, a mio parere. In primo luogo, è stato soppresso l'assurdo obbligo di scegliere in via preliminare l'area funzionale, giudicante o requirente, cui essere assegnati dopo l'espletamento del concorso. Una piccola traccia di questo grande contenuto - secondo l'allora maggioranza - era rinvenibile nell'ultimo emendamento che il collega Valentino ci ha chiesto di votare e che è stato respinto. Abbiamo ritenuto che questa opzione preventiva non fosse assolutamente compatibile con l'impianto complessivo previsto dalla Costituzione. In secondo luogo, abbiamo cancellato - e nessuno l'ha detto - nell'ambito delle prove orali il contestatissimo *test* psicoattitudinale. Su questi due punti, che sono stati gli argomenti sui quali l'Associazione nazionale magistrati ha fatto una campagna durissima nella scorsa legislatura (e penso che queste cose le dirà anche il collega Centaro che interverrà dopo di me), ho l'impressione che qualcuno abbia la memoria corta, perché se l'ANM avesse la capacità di conservare una nitida memoria del recente passato, probabilmente apprezzerebbe molto di più il presente e non minaccerebbe azioni - come dire - "ritorsive" ‑ tra virgolette ‑ il futuro. Come affermava poco fa il collega della Lega, ci si accusa di avere subito la dettatura del provvedimento da parte dell'Associazione nazionale magistrati, poi da altri subiamo l'accusa di essere contestati dall'Associazione nazionale magistrati:

convinta, consapevole di quello che era e di quello che invece è lo scenario che si prefigura. Per fortuna non tutti i magistrati la pensano nello stesso modo: per esempio c'è una intervista a Pierluigi Vigna sul «Corriere della Sera» in cui in qualche modo dà conto

Il nuovo concorso, così come previsto dall'articolo 1, si configura come una prova di secondo grado, che dovrebbe evitare così tutti i problemi che sono sempre nati con l'obbligo di snellire il quadro dei partecipanti con la preselezione, con tre prove scritte. Abbiamo eliminato la previsione di un quarto elaborato pratico proprio recependo delle indicazioni e degli emendamenti che venivano anche dall'opposizione. Tra le altre novità di rilievo che è giusto lasciare agli atti - e mi avvio a concludere, perché sono il contenuto preciso dell'articolo 1 - c'è da ricordare sicuramente la modifica circa la composizione della commissione per l'accesso in magistratura. Abbiamo lavorato molto su questa parte del provvedimento, abbiamo contemperato diverse esigenze, abbiamo accolto moltissimi emendamenti dell'opposizione, alcuni proprio in questa materia anche in Aula, e su questo voglio dire - per essere equanime - che per la prima volta nella commissione di concorso per l'accesso in magistratura sono presenti gli avvocati accanto ai docenti universitari. Come ho detto poc'anzi per l'ANM, il dispiacere è che anche in questo caso, pur avendo introdotto una novità assoluta, che poi coincide con la filosofia complessiva di tutto il provvedimento, dobbiamo riscontrare che anche gli avvocati sono in agitazione. Probabilmente se riscontriamo, da una parte, l'agitazione degli avvocati, dall'altra, quella dei magistrati possiamo essere consapevoli che, fino a questo punto, il provvedimento va in un'unica direzione: quella di recuperare l'efficienza della giustizia, senza guardare a nessuna categoria se non a quella

contro l'articolo 1 perché, in realtà, il problema non era quello indicato dal collega Manzione, cioè un elenco di negatività, di incongruenze e di prove che appesantivano il concorso. Il vero problema era quello di prevedere un concorso che innovasse e modernizzasse l'accesso in magistratura attraverso una selezione diversa e che, soprattutto, costituisse un punto di partenza ai fini della distinzione delle funzioni che, tra l'altro, compare in maniera assolutamente esplicita nel programma dell'Unione. Si parla di distinzione accentuata delle funzioni, ma in realtà così non avviene perché, a differenza del testo della riforma Castelli in cui già dal concorso si ipotizzava una divaricazione, attraverso una manifestazione di volontà del concorrente nei confronti dell'una o dell'altra funzione, in questo modello di concorso tutto ciò non avviene. C'è un pasticcio - di cui parleremo in seguito - per quanto attiene alla distinzione delle funzioni e noi riteniamo che già dal concorso si debba delineare

tra le categorie elencate è scomparsa quella dei rappresentanti delle Forze armate dello Stato, con una certa incongruenza, perché se vengono ammessi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con qualifica dirigenziale - e tali sono, in realtà, anche coloro che militano nelle Forze armate dello Stato raggiunto un certo livello o grado che viene equiparato alla qualifica dirigenziale - ci si rende conto di come poi alla fine ciò che è stato tolto esplicitamente rientri dalla finestra; però, l'averlo tolto ha avuto come significato una sfiducia nei confronti dei rappresentanti di queste categorie. La stessa problematica relativa all'anzianità maturata in diversi rami dell'amministrazione e le stesse materie indicate danno conto di un concorso rimasto vecchio.

meglio il presente dell'economia. Lo stesso dicasi per le problematiche relative alle lingue straniere. Si introduce finalmente un timido accenno alle lingue straniere, però si rimane sempre, tutto sommato, nell'ambito dell'Unione Europea. Nulla vietava che anche la lingua araba vi potesse entrare, considerato che l'Italia è zona di frontiera e si confronta con problematiche (tra cui l'immigrazione, la presenza di gruppi

come è loro abitudine d'altra parte. Infatti, ricordo che anche nella XIII legislatura, nell'ambito della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale e nella riforma costituzionale dell'articolo 111, dell'articolo 111, con posizioni di maggioranza e minoranza identiche a quelle attuali, la magistratura cominciò ad agitare spauracchi dicendo che il Parlamento stava per abrogare per legge la mafia, la lotta alla mafia e quant'altro: non è avvenuto nulla di tutto ciò. allora rendere conto che, nella migliore delle ipotesi, c'è una ritrosia culturale nei confronti del nuovo, nella più realistica delle ipotesi, una assoluta chiusura contro qualsiasi riforma che possa comportare un mutamento dello *status* *quo,* un venir meno di incrostazioni di potere e di controllo, anche fin dall'accesso al concorso in magistratura, utile a far vivere le correnti, utile a quella autoreferenzialità che la magistratura italiana continua sempre ad avere e che la porterà inevitabilmente ad una delegittimazione.

un concorso di secondo grado rispetto a quello precedente, ma che nella sostanza non risponde ad una serie di esigenze fortemente avvertite rispetto ad alcuni temi importanti. La selezione va effettuata tra soggetti di assoluta qualità e questa qualità deve emergere sulla base delle attività precedenti, delle pregresse esperienze, delle attività svolte: non vi è manifestata un'esigenza del genere. Le funzioni che si vanno ad affrontare dopo aver vinto il concorso certamente non possono essere opportunamente tutelate da quel simulacro di tirocinio che si svolge. svolge. Non vi è un tirocinio adeguato. Eppure di lì a poco, questi giovani, che non hanno una particolare esperienza, non hanno maturato nella vita di relazione contatti utili ad un esame più compiuto e più sereno delle complesse realtà con le quali si confronteranno, assumeranno un ruolo di grande responsabilità: saranno magistrati, decideranno della libertà delle persone e dei loro patrimoni: come qualcuno ha detto, decideranno delle anime dei soggetti dei quali dovranno occuparsi. Francamente, avevo confidato che nel corso della discussione in Aula queste esigenze sarebbero state avvertite maggiormente e che vi sarebbe stato un dialogo più aperto; invece no: ci troviamo di fronte agli schemi tradizionali, le nostre proposte vengono sistematicamente rigettate, non si discute. Ma tra i colleghi della maggioranza non c'è alcuno che su questo tema così sensibile, significativo ed importante,

dalla contrapposizione tradizionale degli schieramenti: qui si tratta delle garanzie dei cittadini. Stiamo discutendo delle garanzie dei cittadini e degli uomini che di queste garanzie si debbono rendere interpreti e non si leva una voce a proporre una soluzione? È stato il È stato il compito del relatore, certamente apprezzabile. Egli ha valutato anche con favore talune proposte che sono giunte dall'opposizione; però, devo dire che tutti momenti residuali rispetto ad un'esigenza così vasta che qui, nel dibattito in Aula, avrebbe potuto rivelare

sede che le funzioni più avvertite dall'opinione pubblica debbono trovare i loro interpreti e i loro adeguati propositori. Così non è stato e quindi verrà votato un documento pallido, un documento non particolarmente

contribuirà a fare un passo avanti. Bene, non avete reso un buon servizio al Paese.

Presidente, il Gruppo UDC voterà contro l'articolo 1. Le ragioni le indicherò con maggiore precisione in riferimento all'articolo 2 se, come temo, la bocciatura degli emendamenti essenziali che abbiamo presentato,

che ritengo assolutamente inadeguata per risolvere i problemi della giustizia italiana. c'era un bellissimo film orientale, «Rashomon», nel quale lo stesso episodio veniva raccontato da persone diverse e ciascuno vedeva una realtà completamente diversa. In questo caso non so se stia accadendo la stessa cosa o se semplicemente stiamo facendo il gioco delle parti, ma l'intervento del senatore Manzione, francamente, è abbastanza sconcertante. Ha dipinto una realtà che io, almeno personalmente, non ho assolutamente letto, e cioè quella di una maggioranza che ha dialogato con l'opposizione, che ha aperto alle ragioni dell'opposizione, ha accolto emendamenti dell'opposizione. Non è stato assolutamente così. Una cosa è vera: il clima che si respira in Aula è molto diverso da quello che si respirava quando veniva discussa la cosiddetta riforma

L'articolo 1 è quello sul quale sicuramente siamo meno distanti, perché la sua *ratio* fondamentale è quella che avevamo posto e che questa maggioranza ha accettato.

la maggioranza - bontà sua - ha accettato qualche piccolo emendamento tecnico, ma questo credo sia inevitabile, atteso che abbiamo cercato di migliorare ciò che era comunque migliorabile. Quanto ai tempi, vorrei ribadire quanto abbiamo già rilevato e continueremo a rilevare nel corso di questo dibattito, ossia l'assurdità delle argomentazioni portate avanti dall'Unione.

sono molto più determinati di noi quando intendono portare avanti un qualche provvedimento. Che la chiusura sia totale, però, lo dimostra il fatto che sui dati fondamentali non vi sia stata alcuna modifica di questa norma.

Presidente, stiamo per esprimere un voto importante sull'articolo 1. 1. Già questa mattina ho segnalato al segretario del Consiglio di Presidenza, il collega Barbato, e poi anche agli uffici,

già questo sarebbe un vantaggio sia per la maggioranza che per l'opposizione (perché così chi intende farlo lo fa e chi non intende farlo non lo fa). Meglio sarebbe assegnare i posti a ciascun Gruppo;

alla presenza amministrativa ed evitare la sanzione per l'assenza, anche quando non si è materialmente presenti e votanti, reca un danno economico alle casse del Senato e fa venire meno la funzione stessa della sanzione, che rappresenta più che altro un modo per invogliare i colleghi ad essere presenti.

Grazie, Presidente. Soffermo la mia attenzione e richiamo quella del relatore e del Governo in particolare sull'emendamento 2.201, che interviene sul primo capoverso dell'articolo 11 richiamato nel testo. Siamo al comma 2 dell'articolo 2. Recita la disposizione, in tema di valutazione della professionalità, che tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio, a decorrere dalla data della nomina:

Non ho fatto, signor Presidente, due esempi a caso. Ho parlato di due magistrati, uguali a tutti i magistrati, che hanno, tuttavia, rispetto a tutti i magistrati una peculiarità: sono componenti di diritto del Consiglio superiore della magistratura. L'emendamento che propongo limita le valutazioni di professionalità a tutti i magistrati che sono pervenuti a subire o comunque a sostenere la settima valutazione e quindi non a quelli di maggiore anzianità di età e di età nella magistratura. Quindi, di fatto, viene ad escludere quantomeno questi due soggetti. È opportuno che questi due soggetti vengano esclusi dalla valutazione di professionalità, sembrandomi incongruo che il Consiglio superiore della magistratura, cui è deputata la valutazione di professionalità dei magistrati, possa valutare suoi componenti. Non si capisce che cosa dovrebbero fare il procuratore generale e il primo presidente della Cassazione nel momento in cui scatterà anche nei loro confronti la scadenza ciclica della valutazione di professionalità. Lo stesso problema, peraltro, si pone in qualche maniera per tutti gli altri magistrati che sono componenti del Consiglio superiore in quanto eletti. La legge non dice da nessuna parte che vengono sospese le valutazioni di professionalità nei confronti di questi magistrati e quindi si deve supporre che anch'essi vi siano sottoposti. Richiamo la sua attenzione, signor Presidente, e quella del Governo e del relatore, sul fatto

del Consiglio superiore della magistratura sono tecnicamente magistrati fuori ruolo). Pertanto, sollecito l'approvazione di questo che non ha carattere di assoluta risolutività. Credo infatti che il problema del trattamento dei magistrati componenti di diritto e componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura debba essere affrontato nelle nostre Camere

ma credo che dopo trent'anni di carriera, perché di questo stiamo parlando, si possa anche esonerare senza danno il magistrato da valutazioni di professionalità ulteriori. In tal modo, si consegue il risultato indotto di cui ho parlato di non creare imbarazzanti ragioni di incompatibilità all'interno del Consiglio superiore della magistratura, facilitandone quindi il funzionamento.

è ovvio, e l'abbiamo detto mille volte, che sotto il profilo istituzionale, regolamentare e costituzionale i senatori a vita hanno tutto il diritto di votare, ma è altrettanto ovvio che, dal punto di vista della volontà democratica, anche oggi questo provvedimento è passato non per il voto degli espressi dalla volontà popolare ma perché un senatore a vita ha dato il voto decisivo affinché questo provvedimento passasse. Signor Presidente, mi rendo conto di dire delle parole gravi, ma dobbiamo cominciare a pensare quale sia il titolo di rappresentatività di questa Camera, se veramente sta rappresentando il voto popolare o se, da un punto di vista sostanziale, dobbiamo pensare che essa è illegittima. È un punto sul quale dobbiamo meditare attentamente, perché non è possibile far passare provvedimenti di questa importanza con un voto che si sa *a* *priori* essere in qualche modo inquinato da brogli o da altri elementi che non rispettano la volontà popolare. Questo dobbiamo dirlo perché dobbiamo tener conto di tali questioni, dobbiamo

Senatore Garraffa, si sono già iscritti a parlare due esponenti del suo Gruppo. Lei non ha titolo, quando vuole, per il volume della sua voce, di intervenire così!

E comunque, vedo che lei non perde occasione per dimostrare il suo grande acume e la sua grande intelligenza; perché gli interventi non li fa al microfono, anziché farli sempre fuori? Non abbiamo mai il piacere di sentire gli alati interventi del collega al microfono; invece interviene sempre fuori sacco. Ma intervenga al microfono, dica la sua, ci faccia partecipi della sua grande e profonda cultura e intelligenza!

Presidente, le parole pronunciate in quest'Aula dal senatore Castelli sono le più gravi che possono ascoltarsi da un parlamentare. Egli ha in questo minuto - dovrebbe investire ciascuno di voi, colleghi - contestato la legittimità di quest'Aula e lo ha fatto sulla base di alcune considerazioni che vorrei sottoporre a rapidissima verifica. La prima è che quest'Aula è composta da soggetti che sono stati eletti sulla base di brogli elettorali. È un'accusa che conosciamo dall'inizio della legislatura; la conosciamo per quanto riguarda i colleghi che sono stati eletti in questo Paese sul territorio nazionale e la Giunta delle elezioni ha provveduto, con un lavoro attentissimo, a sbugiardare questa menzogna! E più a fondo andremo, più menzogna apparirà! Per quanto concerne i brogli per gli italiani eletti all'estero, è l'Ulivo che chiede formalmente un dibattito pubblico su questa mistificazione e su questa macchinazione che non riguarda né l'Ulivo né la maggioranza; riguarda, colleghi, e dovrebbe preoccuparvi, esattamente tutti Vorrei ancora ricordare ai colleghi che sono così attenti in questa legislatura che nella scorsa legislatura ben 11 deputati eletti restarono fuori dalla Camera, che mai raggiunse il suo numero perfetto, per un atto di protervia e di arroganza che nella Giunta delle elezioni impedì che 11 eletti sedessero e consentì che un non eletto prendesse il posto per tutta la legislatura del collega Faggiano,

Per quanto riguarda il voto del senatore Andreotti, l'argomento è frusto e inutile e ancora una volta - io ritengo - assolutamente offensivo della lettera della Costituzione, che dice il Senato è composto da senatori eletti e da senatori a vita e non opera nessuna distinzione tra le funzioni, le attribuzioni, i poteri e i doveri degli uni e degli altri.

*(FI)*. Signor Presidente, quello che è successo poc'anzi in occasione dell'approvazione dell'articolo 1 di questa riforma è un fatto che ha una rilevanza politica. Non mi aggiungo al coro di coloro i quali sostengono che il voto dei senatori a vita è un voto affievolito e privo di valenza parlamentare (è la Costituzione che lo prevede e nessuno di noi ha messo in dubbio il significato, l'attuazione la validità dei nostri princìpi costituzionali), ma nell'attuale legislatura viviamo un dato anomalo: in quest'Aula del Parlamento, questa maggioranza questa maggioranza sopravvive grazie al voto determinante, spesso e volentieri, com'è successo poc'anzi, dei senatori a vita, questo è il dato politico. *(Applausi Conosco, stimo e rispetto la collega Finocchiaro e ho imparato a capire che quando i suoi toni pacati, che le fanno onore, vengono vengono sostituiti dai toni dell'aggressività, ciò nasconde uno stato di difficoltà politica della collega. Ha la mia solidarietà, nella difficoltà politica, ma le cose stanno così. FI).* Quello che è successo poc'anzi va analizzato, non va contestato sotto il profilo costituzionale, ma quello che dice il collega Castelli è importante e a questo noi ci aggiungiamo: il senatore a vita Giulio Andreotti, che rispettiamo (è stato il senatore Andreotti come poteva essere il senatore Colombo, il senatore Ciampi e altri), privo di un mandato elettorale, privo di una rappresentatività dei cittadini, si è assunto la responsabilità di fare in modo che questa riforma probabilmente entri in vigore in assenza di un mandato rappresentativo dei cittadini. I cittadini italiani, quindi, vedranno arrivare, probabilmente entro la fine di luglio, una controriforma rispetto a una legge che era stata approvata da un Parlamento sovrano, con una maggioranza elettorale rappresentativa dei cittadini che poi è stata congelata da un Governo che non ha una maggioranza in Senato, il quale poi non soltanto la sospende ma addirittura impone una controriforma che svuota una riforma legittimamente votata. FI).* Le notizie di queste ore, colleghi della maggioranza, sui presunti - mi innamoro della parola presunti - brogli elettorali per i parlamentari eletti all'estero gettano un'ombra di ulteriore preoccupazione, di ulteriore dubbio sulla legittimità di quest'Aula; non dico che quest'Aula è illegittima, ma che vi sono ombre che si accentuano sempre di più quando assistiamo alla proiezione di video con mani che compilano schede inviate alle case dai patronati o da altri, per realizzare per la prima volta un sistema di voto che andava tutto monitorato e analizzato, in assenza della possibilità di una verifica della legittimità dei voti all'estero e in assenza anche della possibilità di un'operazione di controllo di tutte le schede dei voti espressi alla Camera. Signor Presidente, se la maggioranza desse una mano realmente affinché si facesse chiarezza,

su questo testo importante, assumendoci la responsabilità di una opposizione che è consapevole di non essere più minoranza in quest'Aula e di non essere più minoranza nel Paese, perché abbiamo un'ambizione: quella di dimostrare agli italiani con il nostro comportamento, con le nostre denunzie, di essere maggioranza nel Paese e futura maggioranza di Governo.

innanzi tutto voglio associarmi alla richiesta che qui è stata avanzata di una discussione pubblica sui risultati delle elezioni, per tutte le cose che si sentono dire e che sono manifestamente prive di ogni fondamento. BALDASSARRI l'argomento che ha sollevato il senatore Schifani è francamente frusto: abbiamo già affrontato la questione dei senatori a vita, è inutile tornarci sopra, hanno piena legittimità di voto in quest'Aula, votano come hanno diritto di fare, e nessuno può sollevare questo problema. Terza questione: si chiamano sicofanti, senatore Castelli, nell'antico linguaggio della democrazia di Atene, coloro che raccontano dei fichi. Nella Repubblica di Atene i fichi costituivano un tesoro che veniva custodito, appunto, dalla Repubblica come uno strumento per sopportare gli assedi (i fichi sono notoriamente dei frutti dotati di grande potere nutritivo) e venivano pertanto tenuti in celle riservate, segrete. Si chiamavano dunque sicofanti coloro che raccontavano dove si trovavano i fichi, cioè che raccontavano ai possibili ladri dove andare a derubare il tesoro della Repubblica.

da quella parte per sapere chi ruba sul voto, perché lì, in quei banchi, ci sono moltissimi che rubano sul voto e fanno poi quei risultati che abbiamo visto. Quarto ed ultimo argomento: la senatrice Pisa, che è qui dietro di me e può poi testimoniare, risulta tra quei senatori che non hanno partecipato al voto che ha portato al risultato Ora, la senatrice ha partecipato al voto: lei lo dichiara, io e il senatore Iovene, che siamo seduti davanti a lei abbiamo visto il voto della senatrice Pisa, espresso in senso favorevole; ciò nonostante, la macchina non lo ha registrato. cose, i voti non sarebbero 152 a 151, ma 153 a 151 e molto del castello di carte che qui è stato sollevato

Sul problema dei voti espressi, un conto è che un senatore abbia espresso il voto, e ovviamente non ho alcun problema a ritenere che sia così, altro conto è che il voto sia stato espresso al momento della chiusura della votazione. infatti toccano i tasti per leggere il risultato sul *monitor*: questa operazione, se si sbaglia, determina la cancellazione del voto se viene effettuata prima della chiusura, e lo dico anche in riferimento ad

avrei evitato di parlare se la collega Finocchiaro non avesse ricordato una vicenda che riguarda la Camera dei deputati nella precedente legislatura, accusando in maniera del tutto generica per il fatto che 11 deputati non poterono entrare alla Camera dei deputati. Non vorrei che restasse il dubbio da parte di alcuni che questi 11 deputati che dovevano entrare fossero tutti del centro-sinistra, perché non è così:

dei senatori a vita. L'ho detto fin dal primo momento e lo voglio confermare anche in questa occasione: i senatori a vita hanno gli stessi diritti e doveri di tutti noi e non è che diventino bravi quando votano per il centro-destra mentre esprimano un voto illegittimo quando votano per il centro-sinistra; sarebbe uno sbaglio ragionare in questi termini, perché hanno il diritto di votare come meglio credono. In questa circostanza, però, trattandosi di un voto sulla magistratura, rispetto al voto del senatore a vita che ha determinato la vittoria da una parte

ha mandato in onda una intervista di un Ministro in carica che polemizzava contro questo provvedimento. Dovete riuscire a chiarire al vostro interno se questo ordinamento debba passare o no: è un problema che deve essere risolto al vostro interno. Noi certamente lo avversiamo, perché vogliamo che

è un atto politico. Ci mancava, in questo anno di governo, lo sciopero della magistratura, così tutte le categorie produttive del Paese avranno scioperato contro di voi; mancava la magistratura, ma ora si assisterà anche allo sciopero Dovete prendere atto di questo e non potete soffermarvi sul perché nella precedente legislatura non sono entrati 11 deputati, perché non è questo l'argomento. Chiarite, ripeto, i problemi politici che avete

o daranno una mano per il futuro a non costruire castelli in aria. Intanto ringrazio il presidente Matteoli, perché ha riportato nel clima giusto la discussione che deve esserci tra di noi.

dopo un anno di discussioni sulle stesse questioni, pare che non ci si ricordi che la nostra maggioranza è di due voti e che quindi, teoricamente, su ogni provvedimento potremmo registrare solo e soltanto due voti di maggioranza. Se questo ritornello lo dobbiamo sentire fino alla fine, non facciamo un buon servizio ai lavori. Vi sono Parlamenti di altre Repubbliche in cui per un voto l'intera legislatura si è portata a compimento fino al suo normale esaurimento. esaurimento. Quando si intende invece attaccare ripetutamente ed ossessivamente su questo aspetto - e, ripeto, ero tra i non partecipanti al voto, non perché non condivida il provvedimento del ministro Mastella, ma perché ero ad una conferenza stampa insieme con altri parlamentari presenti, perciò chiarisco e sto intervenendo in questo senso - mi pare non si possa andare avanti all'infinito senza ricordarsi che la nostra è una maggioranza per due voti, quindi senza che desti scandalo se su un articolo, un provvedimento o un singolo atto vi siano uno o due voti di maggioranza: è successo e succederà ancora.

per fare presente alla presidente Finocchiaro che quanto lei ha detto è quantomeno impreciso. Capisco la foga che ha portato la collega ad alcune considerazioni un po' demagogiche: è il nervosismo del magistrato in aspettativa, oggi presidente di un Gruppo parlamentare, nella discussione di questo provvedimento. Non si può però affermare che ci sia stata una campagna di menzogne sui brogli elettorali e che questa campagna sia stata sbugiardata, per almeno una semplice ragione: che, intanto, il lavoro di accertamento sul voto degli italiani in Italia si sta svolgendo e non è ancora giunto a nessuna conclusione, quindi non c'è nessuno sbugiardamento di alcuna menzogna ai fini delle nostre acquisizioni. Per quanto riguarda poi il voto degli italiani all'estero, è fatto conclamato tra i membri della Giunta - ma penso anche di tutto il Senato e da tutto il Paese - che la maggior parte dei verbali che ci sono giunti dalle sezioni di scrutinio del voto degli italiani all'estero sono in bianco, non sono compilati ed è impossibile compilarli, quindi abbiamo avuto sei colleghi eletti sulla base di

senza citare quanto ha pubblicato Deaglio su "Diario". Il problema, cara collega Finocchiaro, non è la velenosa campagna che proviene dal vostro velenoso interno

di legittimità del voto, ma il fatto che normalmente sul piano politico la maggioranza considera quello come il suo esercito di riserva e si impegna a mobilitarlo come un partito della coalizione nei momenti difficili, e si assistono i senatori a vita sinanche nelle loro funzioni basilari, curandoli come i badanti curano degli anziani non in grado di essere autosufficienti. Questa non è libertà di determinazione, questa è prevaricazione

prendano atto che stanno prevaricando sulla base di una serie di fatti e di incertezze in questa fase la vita parlamentare e il Paese e che da parte dell'attuale opposizione era giunta loro una mano per condurre le istituzioni nell'alveo di un rapporto democratico che loro hanno rifiutato e morso, e tutti gli abusi che stanno commettendo non possono che chiamarsi tali. *(Applausi

non solo sui senatori a vita. Ricordo che un senatore a vita è stato candidato alla presidenza del Senato, perciò legittimamente, nel pieno delle sue funzioni. Ricordo, inoltre, che il Governo, forse, è stato sconfitto anche per il voto dei senatori a vita in alcuni passaggi e, ancora di più, ricordo che, forse sbagliando, quest'Aula ha deciso di votare le dimissioni di un senatore a vita. Dico "forse sbagliando" perché non era proprio, ma con ciò sottintendendo che il senatore a vita è esattamente come qualsiasi altro senatore eletto.

fatta - su chi vota e non c'è: in un'altra votazione ha votato un senatore del centro-destra che, secondo prove documentate, presiedeva in un altro luogo un'altra riunione. Ma questo attiene al Presidente e ai segretari che controllano l'andamento del voto. È stata qui sollevata, invece, una questione più grave che attiene alla legittimità della votazione ed è stata posta anche nell'ultimo intervento. È più grave per chi, come me,

che i vostri Ministri abbiano garantito al Paese una libera e democratica elezione. Signor Presidente, anche l'UDC vorrebbe che fosse conclusa la valutazione sulle due questioni di fondo sulle quali si è intrattenuta la collega Finocchiaro. Non vi è mai stato alcun dubbio da parte del centro-destra, e neanche ovviamente da parte del collega Castelli, sulla legittimità del Senato in quanto tale come organo rappresentativo dell'ordinamento costituzionale italiano. Le deliberazioni assunte anche con il voto determinante dei colleghi senatori a vita sono valide e nessuno lo ha messo in dubbio. La questione politica che il Capo dello Stato ha indicato o ha fatto ritenere indicata quando il Governo Prodi si è dimesso è un'altra e invito i colleghi del centro-sinistra a considerarla anche in riferimento all'ultimo voto: occorre che la maggioranza, politicamente, non legittimamente, sia autosufficiente rispetto ai senatori a vita. Si è detto che devono essere 158 i senatori della maggioranza eletti

concorre a far venir meno quella regola politica - non di legittimità - del voto sulla quale noi siamo particolarmente sensibili. Sappiamo che la maggioranza è tale in quest'Aula per soli due voti, ma deve essere capace di reggere il confronto parlamentare. Se non lo regge non è più maggioranza politica, non legittima. I senatori a vita devono legittimamente aggiungersi al voto dei 158 al voto dei 158 o, se sono meno di 158, ai voti politici. In quest'Aula i voti politici non erano in maggioranza rispetto all'opposizione. Questo è il dato politico che fa emergere l'ultima votazione.

attento ad altre cose in questo momento essendo il capogruppo del Gruppo che fa capo al ministro Di Pietro, che notoriamente non ama il ministro Mastella. Vorrei che il senatore Formisano fosse più presente in quest'Aula: per evitare il sospetto, caro Formisano!

desidero scusarmi con il mio Gruppo e con tutti i colleghi, perché ho letto che non ero presente al momento della votazione. Sono dispiaciuto, perché credo che tra le poche qualità di cui possa vantarmi ci siano quelle della diligenza e anche della coerenza e non avrei mancato in un momento delicato. Non avevo la visione complessiva dei problemi. Devo confessare che soffrono d'asma ogni tanto ho bisogno di allontanarmi e non avevo in tasca quel che sono andato a recuperare poco fa, che mi serve anche per poter parlare con maggiore serenità. *(Il senatore perché so che in queste situazioni si verifica una sorta di legittima suspicione*,* come mi è parso anche poco fa di capire, circa le presenze e le assenze. Siamo parlamentari, però abbiamo, anche nella funzione di rappresentanza, gli stessi limiti e talvolta gli stessi acciacchi che hanno coloro che ci mandano qua. Perciò chiedo scusa e vorrei che fosse considerato quel che ho detto una giustificazione fisica e politica, e vi ringrazio per l'attenzione e il rispetto con i quali seguite sempre le mie parole.

linearità in questa discussione. Il senatore Formisano, illustrando i motivi per i quali non ha partecipato ai lavori dell'Aula, ha dichiarato che

Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei dire che quando si è cominciato il lavoro sui risultati elettorali nessuno ha mai messo in discussione, né nella maggioranza, né nell'opposizione, la regolarità del voto per il Senato in Italia. Questo problema non si è mai posto e il risultato, in Italia, era perfettamente regolare, tant'è che ha vinto la Casa delle Libertà, ottenendo oltre 200.000 voti e due senatori in più. Il problema si è posto quando, in conseguenza del voto estero, è stata ribaltata la maggioranza elettorale che ha vinto le elezioni in Italia e quindi tale problema, nonostante quello che dice la senatrice Finocchiaro, diventa serio, molto serio. Quando si è trattato di controllare i voti per il Senato in Italia, questo non è avvenuto perché l'ha richiesto la maggioranza o l'opposizione o perché l'ha richiesto il presidente Berlusconi, le cui osservazioni si riferivano sempre ai 24.000 voti in più alla Camera e al fatto che, mentre al Senato la CDL aveva vinto di oltre 200.000 voti, alla Camera c'era stato un risultato diverso. Il conteggio, al Senato, Regione per Regione, si è fatto in conseguenza della circostanza che il noto Deaglio ha sostenuto che si era verificato un falso elettorale, quindi noi siamo stati «costretti», per difendere l'istituzione Senato, a fare un controllo che, di fatto, ha dimostrato la verità del risultato elettorale. Ha ragione la collega Finocchiaro: in Italia al Senato ha vinto la Casa delle Libertà e quindi il controllo è perfettamente regolare. Come si è posto allora il problema? Si è posto, in conseguenza della decisione presa da noi al Senato, per la Camera: sarebbe stato naturale, se davvero la maggioranza crede nella correttezza del processo democratico, che alla Camera avessero proceduto immediatamente al riconteggio delle schede perché, fatte le simulazioni, non bisogna mai dimenticare che 24.000 voti di differenza credo che corrispondano a quattro voti in un Comune di 5.000 abitanti, più o meno. Cioè, in qualunque Comune, da qualunque parte, di fronte ad uno scarto così esiguo, si sarebbe proceduto al riconteggio delle schede. Orbene, alla Camera quel conteggio è stato avviato in conseguenza della delibera presa al Senato, perché sarebbe stato veramente grave che il presidente Bertinotti, una volta che al Senato si era deciso di ricontare le schede, non avesse proceduto in tal senso alla Camera.

a causa di una precedente delibera, al controllo puntuale, specifico e preciso, dei voti nella circoscrizione estero. Per questo, di fronte a ciò che è avvenuto, di fronte alla gravità del video, di fronte alla circostanza che quel video è stato pubblicato su «la Repubblica.it» e che la denuncia parte in conseguenza di quanto dichiarato da un appartenente all'Udeur che è un partito dell'Unione, perché tutti quanti, con l'approvazione della maggioranza, non procediamo subito in Giunta al controllo del risultato delle circoscrizioni estere? Infatti soltanto alla luce di questo passaggio noi sapremo se la maggioranza che c'è al Senato se la maggioranza che c'è al Senato corrisponde davvero alla scelta degli elettori. Concludo dicendo che è vero che il voto dei senatori a vita è un voto come tutti gli altri, solo che il problema non è il voto il voto ma il suo effetto. Già Napolitano, il presidente della Repubblica, ha spiegato che non può esistere, in un Paese democratico, una maggioranza politica che si regge sul voto dei senatori a vita, non fosse altro perché sono stati scelti per meriti particolari che danno lustro alla patria e tutta una serie di considerazioni che non hanno nulla a che vedere con la politica. Certamente, constatare che, normalmente, un Governo si salva con il voto dei senatori a vita è qualcosa che, dal punto di vista del processo democratico, quantomeno lascia molti dubbi.

formulare solo tre considerazioni velocissime: occorre effettivamente fissare un dibattito su questa materia, che è complicata assai; così come occorre un dibattito complessivo su come viene esercitata in questo Senato l'autodichia, la capacità, riconosciuta alle Camere dalla Costituzione, di essere giudici di se stessi. Questo, signor Presidente, perché nelle Aule assistiamo ad un dibattito nel quale maggioranza ed opposizione si scambiano reciproche accuse, fermo restando che mercoledì abbiamo assistito ad un dibattito diverso, nel quale una parte della maggioranza e tutta l'opposizione hanno raggiunto un accordo - che ho definito ignobile e che ribadisco essere tale - in forza del quale, per sostituire il collega Vernetti, che si era dimesso,

che, secondo le norme vigenti, spettava alla Commissione elettorale regionale del Piemonte. La Giunta si è appropriata di un diritto che non le spettava e ha indicato il senatore Bobba, che poi ha optato, escludendo l'avente titolo e privilegiando il collega il collega Ria. In questo modo, però, al di là di tale meccanismo, che ha violato la legittimità del *plenum*, dal mio punto di vista, ha creata un *vulnus* ancora più grave: la legge, infatti, prevede che gli aventi diritto possano chiedere alla Giunta delle elezioni di valutare il comportamento di chi propone l'elezione.

sul proprio comportamento: quindi, un *vulnus* ed una violazione enormi. In secondo luogo, si parla di questo video pubblicato da «La Repubblica»: ma dimentichiamo - e lo fa soprattutto il presidente Nania - che più volte ho messo agli atti che era necessario procedere alla verifica per la circoscrizione estero.

ossia la questione della Rosa nel Pugno e degli altri ricorrenti che pretendevano soltanto una cosa, che venisse data loro una risposta. La Giunta, all'unanimità, con una serie di situazioni di incompatibilità mostruose, sostanzialmente sta denegando giustizia: ecco perché, a monte di tutto, occorrerà effettuare una riflessione sulla capacità di questa Camera di conservare al proprio interno il potere dell'autodichia che pretenderebbe esistere il rispetto delle istituzioni, il governo delle istituzioni ed il rispetto di una Costituzione - anche nella sua parte non scritta che pretende un senso di responsabilità per esercitare un potere. Quando quel senso di responsabilità viene meno - come nel caso di specie - vi sarebbe la necessità di

l'articolo sarebbe stato bocciato, così come, se fossi stato di turno io, invece, avrebbe vinto per due voti al posto di uno e così potrà accadere questo pomeriggio, a seconda che vi sia il collega Angius

il 2.101, che è puramente tecnico e riguarda il modo con il quale vengono identificati i tribunali di sorveglianza nel nostro ordinamento.

io che sono stato selezionato per essere un magistrato con funzioni indifferenti, voglio passare dall'attuale sistema della confusione delle funzioni - perché di questo si tratta oggi - al regime della separazione. Quante volte, dopo un certo uno numero di anni nei quali prevale il desiderio di tornare a casa - che non riguarda quindi la funzione svolta - si deve esercitare questo diritto? Riteniamo che, se si tratta della separazione delle funzioni e non della finzione della separazione delle funzioni, occorra un numero di anni che stabiliamo generosamente in dieci, dopo l'immissione nella magistratura, perché si possa una sola volta esercitare questa opzione (o requirente o giudicante). Questo è il senso dell'emendamento proposto. È una questione di fondo, che tende a far capire se stiamo andando dalla confusione delle funzioni alla separazione delle funzioni o se manteniamo il principio della confusione delle funzioni appena attenuato. La Commissione propone non più di quattro volte nell'intera carriera:

Mentre in Commissione avevamo esaminato e respinto un emendamento che tendeva a dire che questa separazione vale soltanto per la materia penale (perché ovviamente tutti capiscono che, se uno ha fatto l'inquirente in materia fallimentare diventare giudice civile in materia fallimentare, non siamo proprio in presenza di nessuna separazione nei confronti dell'indagato) vedo purtroppo con preoccupazione che viene ripresentato in Aula, con autorevolissime firme del collega Massimo Brutti e della collega Magistrelli, un emendamento che reintroduce la finzione della separazione, limitandola solo al penale. allora se per avventura la maggioranza è orientata a trasformare in acqua torbida, ma semplice, la separazione delle funzioni e si prepara a respingere il mio emendamento, che prevede che si passi dalla confusione alla separazione, e ad approvare l'altro emendamento, che rende la separazione delle funzioni ancora più ridicola di quanto non lo sia oggi. In tal senso occorre capire - lo ripeto ancora una volta - che l'assenza di Formisano aveva un valore preciso. Occorre capire che la minaccia di sciopero del 20 luglio significa non approvare l'emendamento della separazione e approvare l'emendamento del senatore Massimo Brutti. Se questo è il caso, allora occorre che la collega Finocchiaro capisca o dica fino in fondo che siamo in presenza di un'ingiunzione, di una minaccia, di una impossibile tesi in base alla quale questo Parlamento non è libero di decidere che cos'è la separazione delle funzioni perché il vertice dell'Associazione nazionale magistrati non vuole neanche che ne parliamo: minaccia lo sciopero solo perché se ne parla. Quando arriveremo all'emendamento 2.138che ho sostenuto, vi sarà un dibattito molto serio e mi auguro molto approfondito e chiederò di intervenire in dichiarazione di voto. I colleghi sappiano che siamo in presenza - è evidente - di un punto fondamentale della riforma: o siamo un'Assemblea libera anche nei confronti dell'Associazione nazionale magistrati o siamo un'Assemblea suddita. Questo era il compito a cui mi auguravo il Governo, con il ministro Mastella, assolvesse; per questo siamo delusi

e capisco l'intesa; oppure, se è la maggioranza che tratta con i magistrati, allora se li tenga, come li ha voluti; si tenga la legge anche con un solo voto, ma capisca che non si è risolto il problema. credo che il senatore D'Onofrio abbia toccato il reale problema di questo ordinamento giudiziario:

quale dei Ministri vincerà la sua partita, quale tipo di ordinamento nella realtà vuole la maggioranza, quanto la maggioranza sia succube dell'Associazione nazionale magistrati. Il che evidentemente mi consente di evitare di far perdere tempo all'Assemblea nell'illustrazione dei miei emendamenti, sì da non poter dare a nessuno la briga di ritenere che sia in atto da parte nostra un atteggiamento di tipo ostruzionistico.

ma in ogni caso lo farei successivamente, quindi non vi sarebbe sotto questo profilo perdita di tempo - di poter riformulare un emendamento. Mi riferisco esattamente all'emendamento 2.103,

mi sembra una proposta ragionevole quella contenuta nell'emendamento 2.202. Nel momento in cui i membri del consiglio giudiziario debbono esprimere un'opinione, che poi avrà delle conseguenze sui magistrati sottoposti alla loro valutazione, credo che l'accesso diretto a documenti che siano pubblici e che rivelino quale ruolo nell'ambito dei vari processi sottoposti alla loro cognizione abbiano svolto quei magistrati, come si siano contenuti, quali esiti abbiano avuto i processi, quale sia stato il rapporto con gli avvocati e con gli altri magistrati, un elemento di valutazione ulteriore che certamente non può turbare alcun equilibrio, anzi, può contribuire a determinare equilibrio. Quindi, raccomando all'Aula perché non mi sembra che stravolga gli assetti della proposta di legge così come formulata ma aggiunga un elemento importante per una maggiore tranquillità nelle determinazioni che in sede di consiglio giudiziario andranno assunte.

si riferisce alla questione già sollevata dal collega D'Onofrio del numero delle volte nelle quali è possibile il passaggio, nel corso della carriera, tra funzione requirente e funzione giudicante. Abbiamo apprezzato in discussione generale il limite che era stato introdotto dalla Commissione relativo alla non possibilità di trasferimento in distretti all'interno della stessa Regione ma vediamo che, in relazione agli ultimi *diktat* dell'Associazione nazionale magistrati, i senatori Formisano

e che quindi il divieto di esercitare funzioni diverse da quelle precedentemente esercitate nell'ambito del distretto della stessa Regione permanga, la possibilità di modificare quattro volte nell'arco della carriera le proprie funzioni, passando per ben quattro volte dalla requirente alla giudicante o viceversa, annulla di fatto ogni barlume di separazione delle funzioni, che pur si è ritenuto di cercare di introdurre in qualche modo in questo provvedimento. Allora, noi proponiamo con l'emendamento

ma, prevederne quattro, come ha fatto la Commissione, significa obiettivamente dichiarare che tutto quello che è stato scritto sulla diversità tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti è una burla e non ha nessuna validità. Significa introdurre un continuo viavai all'interno della carriera di un magistrato tra quelle che sono le due funzioni e, quindi, si vanificherebbe ogni significato della riforma. Per tale ragione confido sulla possibilità di accogliere i nostri emendamenti.

Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 2 si dividono in due categorie; gli emendamenti 2.128 e 2.129 si riferiscono all'anticipata possibilità di arrivo in Cassazione di magistrati più giovani, di fascia cioè inferiore alla quarta, ritenuta congrua ai fini della valutazione per il conferimento delle funzioni di legittimità. Questa ipotesi, che ha avuto un certo favore in Commissione, in realtà, è passata poi monca e si è compiuto una sorta di pasticcio, come è pasticciato l'articolo 2. Perché, in realtà, questa valutazione anticipata doveva essere compiuta attraverso un vero e proprio concorso; ora, nessuno pretende che sia un concorso con esami scritti o esami orali, ma, certamente, oltre ad un concorso per titoli, bisognava almeno aggiungere una prova orale che desse conto della capacità di questi giovani magistrati di poter esercitare adeguatamente le funzioni di legittimità. Diversamente, così come si è previsto in questo momento, abbiamo ipotizzato esclusivamente una quota riservata a magistrati che abbiano valutazione in carriera inferiore a quella ordinariamente indicata ai fini dell'accesso in Cassazione; quindi, a tutta evidenza, una sorta di quota riservata senza un'adeguata valutazione, almeno attraverso un esame orale, dell'accesso in Cassazione. Anche in vicenda assolutamente avversata dall'Associazione nazionale magistrati che vede questo arrivo anticipato *per saltum* di quella che è una graduatoria di anzianità, uno scompaginamento complessivo di quella che è una vicenda di controllo della carriera dei magistrati. E, ugualmente, altro emendamento che riguarda sempre tale vicenda che deve anche ricondurre l'anticipato arrivo in Cassazione attraverso la circostanza che tale possibilità non faccia saltare a piè pari un ruolo di anzianità, che, comunque, deve rimanere integro, e non possa costituire un titolo di merito o privilegiato privilegiato e preferenziale ai fini dell'arrivo in ulteriori funzioni che possono essere funzioni direttive o altro tipo di funzione di merito. Diversamente, infatti, a tutta evidenza, ipotizzeremmo una carriera privilegiata. Gli altri emendamenti riguardano la *vexata quaestio* della distinzione delle funzioni. Dico subito che questi emendamenti si rivolgono per certi versi a problematiche che lo stesso sottosegretario Scotti, in sede di discussione nell'ambito cioè la circostanza che gli uditori, i magistrati nominati di prima funzione, non sempre riescono ad avere funzioni e sedi che possano essere concilianti con le loro aspirazioni professionali o con le loro problematiche e, quindi, hanno necessità di una sorta di possibilità di avvicinamento. Gli emendamenti prevedono la possibilità che dopo i primi dieci anni di esercizio di funzioni e quindi dopo che il magistrato ha avuto la possibilità di pervenire nella sede, nelle funzioni che più gli aggradano, vi possa evidentemente essere massimo due possibilità di mutamento di funzioni nell'arco dell'ulteriore carriera che, badiamo bene, si svolgerà nell'arco di non più di trent'anni, forse meno. meno. Questo tipo di emendamenti, allora, faciliterà certamente questa possibilità nei primi anni, cristallizzerà, com'è giusto che sia, in relazione all'indirizzo all'indirizzo che il magistrato ha ritenuto di dover dare alla propria carriera, le funzioni di questo magistrato attuando, esse sì, una vera e propria distinzione. Altri emendamenti riguardano il *turnover*, la possibilità data ai magistrati di mutare le funzioni nell'ambito dell'intera carriera per non più di quattro volte. Posso dire che, per l'esperienza svolta da magistrato, quattro volte è un numero che non ricorre mai, nell'ambito di un'intera carriera di magistrato, di mutamento da funzioni giudicanti a requirenti o viceversa: succederà al massimo non più di due o tre volte nell'ambito dell'intera carriera questo salto, perché poi alla fine ci si indirizza verso un filone di funzioni e si possono cambiare sedi, si può cambiare

tanto vale cercare di essere più sostanziali, senza far venire meno una possibilità di ritorno di mutamento d'indirizzo, di cambiamento di idea e ipotizzare, creando veramente una distinzione delle funzioni, un cambiamento che se non può essere una sola volta perché sarebbe una cessione eccessiva ad ipotesi di vera e propria distinzione delle funzioni e non ad una sorta di pasticcio come quello ipotizzato dal testo uscito dalla Commissione, ma almeno non più di due o tre volte, che sono dei numeri che corrispondono effettivamente a quelli che sono mediamente i mutamenti che già oggi si verificano nell'ambito della magistratura.

che viene registrato alle ore 12,22, e di cui l'Aula non si può sottrarre dall'essere a conoscenza, e cioè che il ministro Amato, ad un convegno sull'Islam ha dichiarato: «Picchiare le donne è una tradizione siculo-pakistana». Ora, non so cosa il ministro Amato abbia fatto negli ultimi giorni: abbiamo letto sui giornali che è andato a giocare a tennis e che lo ha fatto con Canè, che ha pure vinto, che ha messo un cappellino bianco, ma secondo me ha preso troppo sole, perché commettere un errore del genere, che significa essere richiamati ad una più stretta osservanza dei rapporti tra le Nazioni, e in questo caso non soltanto con le Nazioni ma con l'intero Islam, ed offendere 5 milioni di cittadini italiani, se mi permette, è un eccesso rispetto a cui quest'Aula deve fare voto affinché il ministro Amato chieda scusa immediatamente.

Signor Presidente, sono grato ai colleghi che hanno, nella illustrazione dei loro emendamenti, dedicato una particolare, preventiva attenzione all'emendamento che ho, assieme alla collega Magistrelli, sottoscritto. Vorrei dire per la Presidenza, per l'Aula e per tutti i colleghi, che questo emendamento, cui era sostanzialmente corrispondente l'emendamento presentato dal collega Cusumano, è stato da me, in pieno accordo con la collega Magistrelli e con il collega Cusumano, riformulato in modo tale da renderlo, sotto il profilo tecnico e sotto il profilo della forma linguistica, a nostro giudizio migliore. quindi nel fatto che il nuovo testo da me tempestivamente consegnato alla Presidenza sia stato distribuito a tutti i colleghi. il merito delle osservazioni, in particolare di quelle puntuali proposte dal collega D'Onofrio, voglio dire che noi potremmo qui oggi (e nei mesi scorsi e nella scorsa legislatura avremmo potuto) trovarci di fronte ad una alternativa di modelli organici, coerenti, definiti, circa l'organizzazione della giustizia nel nostro Paese. Io avrei voluto e vorrei che il centro-destra con maggiore coraggio sostenesse, a cominciare dall'esigenza di un mutamento della Costituzione che sarebbe necessario, il principio che ha una sua legittimità e serietà di netta separazione delle carriere. Ciò significa due concorsi, un diverso ordine di responsabilità e perfino un diverso rapporto con il potere politico. Non è ignota agli ordinamenti democratici del mondo contemporaneo questa netta separazione tra le carriere dei giudici e quelle dei pubblici ministeri, e naturalmente essa riguarda l'organizzazione della magistratura che si occupa degli affari penali e che è chiamata ad applicare le norme del diritto penale secondo le regole del codice di procedura penale.

che ha sulle spalle la rappresentanza degli avvocati penalisti ed esprime una cultura giuridica coerente e seria; nonostante, dicevo, la presa di posizione di questa parte dell'avvocatura il centro-destra non ha mai avuto il coraggio di sostenere fino in fondo la separazione delle carriere dei magistrati, con tutte le implicazioni istituzionali e politiche che tale separazione comporta. purtroppo una tradizione nella storia giuridica di questo Paese: tutti i grandi interventi normativi di codificazione o di settore hanno una caratteristica, quella della ricerca di progressivi compromessi con lo stato di cose esistente, con una tradizione consolidata, e naturalmente ciò porta agli aggiustamenti, alle mezze proposte. Ora , io non riconosco alle posizioni qui espresse dal centro-destra la caratteristica di essere ciò che potrebbero e dovrebbero essere, vale a dire proposte rigorosamente alternative all'impianto che invece ispira il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario presentato dal Governo, rimaneggiato dalla Commissione e che noi oggi stiamo discutendo. E allora, la nostra discussione si colloca all'interno di un circuito nel quale tutti, centro-destra e centro-sinistra, riconoscono che la carriera è unica, che molto vi è di comune tra le funzioni giudicanti e quelle requirenti, anche in relazione al dettato del codice di procedura penale del 1989, che tra l'altro fa obbligo al pubblico ministero di raccogliere e valutare adeguatamente tutti gli elementi idonei a scagionare l'indagato e l'imputato. Dunque, di cosa stiamo discutendo? Vi è un'esigenza, diciamo così, di immagine,

non possa da un giorno all'altro uscire dalla porta del suo vecchio ufficio ed andare nell'ufficio che si trova al piano di sotto, diventando il giudice che affronta, sul terreno del processo penale, questioni, casi, controversie, che riguardano le stesse persone, la stessa fetta di popolazione, lo stesso ambiente entro il quale svolgeva fino a ieri le funzioni requirenti penali. È l'esigenza della salvaguardia di una immagine e non è un'esigenza da sottovalutare posto che, a partire dal famoso articolo della legge sulle guarentigie che parlava di prestigio della magistratura, di prestigio dell'ordine giudiziario, tutta l'interpretazione giuridica di questi decenni ha risolto questo concetto del prestigio in un concetto concetto un po' più concreto e verificabile nella vita sociale, che è quello di credibilità del magistrato e che riguarda il rapporto tra il magistrato e l'ambiente entro cui egli opera. Di qui la condivisione larga della utilità di una norma che imponga un determinato tipo di trasferimento - poi dobbiamo concordare come definirlo e il testo in discussione lo fa discussione lo fa - da un ufficio giudiziario ad un altro, proprio perché non vi sia questo *continuum* dall'esercizio della funzione requirente all'esercizio della funzione giudicante sul terreno penale o, viceversa, negli stessi uffici della stessa sede. quindi di fronte ad una norma che va definita e discussa secondo criteri di opportunità e di equilibrio. che in questi anni ho riservato particolare attenzione ad una linea, ad una prospettiva di valutazione del rapporto tra le funzioni e del ruolo dei magistrati che andava in una direzione del tutto opposta e radicalmente alternativa rispetto alla tesi della separazione delle carriere. Secondo me (ma, lo ripeto, faccio una parentesi brevissima, perché si tratta di una mia opinione personale) sarebbe migliore sistema quello che favorisse un passaggio frequente da una funzione all'altra, in modo tale da rendere il pubblico ministero fino in fondo partecipe di una cultura delle prove, di una cultura della giurisdizione e di un punto di vista che è proprio del giudicante, e allo stesso modo in una in una guisa tale da fare svolgere a chi, poi, va ad esercitare le funzioni giudicanti, anche altre esperienze, che lo arricchiscono. Benissimo, questa è una mia opinione personale: è una tendenza, un indirizzo della cultura giuridica che non ha trovato espressione nella legislazione. Ma allora si tratta di trovare un punto di equilibrio per far sì che vi sia una certa distinzione delle funzioni che giovi alla credibilità dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Ma dobbiamo evitare che questa certa distinzione delle funzioni sia dominata (cari colleghi, permettetemi di osservare questo aspetto del dibattito) da una ossessione punitiva nei confronti della magistratura che invade una parte del ceto politico italiano oggi e che è segno di debolezza anzitutto culturale. Non c'è ragione di rappresentare la magistratura come il regno del male o l'associazione nazionale magistrati come una specie di club eversivo. Se qualcuno di noi compie delle scelte in un senso o nell'altro fidatevi, colleghi - lo fa in piena autonomia, perché ha letto qualche libro nella sua vita, perché è convinto che si debba dare alla magistratura italiana e all'esercizio della giurisdizione un assetto equilibrato che giovi alla garanzia dei diritti e all'equilibrio costituzionale. E piantiamola con questa storia dell'ANM che attraverso la figura del Sottosegretario che si insinua nei nostri uffici e nelle nostre Aule ci passa veline o ci impone punti di vista. Non è così. Il Parlamento è sovrano l'associazione nazionale magistrati è una associazione legittima. In tutti i periodi nei quali in Italia ha dominato l'autoritarismo una delle prime cose che è stata fatta è vietare l'associazionismo dei magistrati e disporne lo scioglimento, così come si bruciavano le camere del lavoro e si sopprimeva la libertà sindacale. allora ad un dibattito più sereno ed equilibrato. Valutiamo il contenuto delle proposte, che possiamo accettare o rigettare, in quanto si tratta di proposte che puntano a stabilire un equilibrio, nel quadro di una visione nella quale non vi sono alternative radicali. Se vi fossero, voi dovreste essere i primi ad avere il coraggio di respingere l'intero impianto e ad avanzare qui una proposta di riforma della Costituzione per dividere davvero le carriere dei magistrati.

centro-destra nel corso del dibattito in Commissione era stata sollevata la necessità di inserire questa limitazione nei criteri di valutazione;

2.116 (perché introduce un concorso per titoli ed esami al quale siamo contrari), 2.117

2.217 e 2.218, anche perché non si saprebbe che fine dovrebbe fare il vecchio titolare.

Presidente, concordo con il relatore sul diniego ad una serie di proposte emendative formulate e condivido, da parte del Governo, la richiesta di appellarsi all'Aula per quanto riguarda l'emendamento del che peraltro, lo dico per la storia e la cronaca, in quest'Aula e fuori dell'Aula, a Ministri miei colleghi e ad altri, è statopresentato per primo dal senatore Cusumano del Gruppo dell'Udeur, successivamente dal senatore Brutti, come recita il racconto cronologico, e poi dalla senatrice Magistrelli. Devo aggiungere, con molta obiettività (lo dico con tono fermo e risoluto), che credo che la mia maggioranza debba chiarirsi le idee in ordine all'articolo 2, perché la controversia è più all'interno della maggioranza e un po' meno con l'opposizione, che svolge il proprio ruolo con grande dignità. Spero che uguale dignità e compattezza vi sia anche da parte della maggioranza, della quale faccio parte fino a prova contraria.

la correttezza con cui l'opposizione sta svolgendo il proprio ruolo - di questo non possono che essergli grato - e ha altresì richiamato la

Senatore Caruso, francamente dopo l'appello del Ministro mi sarei aspettato che la richiesta che lei ha fatto, e che mi sembra estremamente fondata sul buonsenso, fosse venuta da un Capogruppo di maggioranza

Presidente, devo dire che la dichiarazione del Ministro può essere considerata a buon diritto un *coup de théâtre* che ci

segnalando che il Ministro evidentemente dà un giudizio assolutamente obiettivo; credo però che la cosa più grave sia la sua seconda dichiarazione. Ora, su tale dichiarazione vorrei che il Ministro fosse più esaustivo:

per quanto riguarda i controlli periodici di professionalità. Si vada a vedere le dichiarazioni rilasciate nei convegni in tutti questi anni: sono riportate addirittura pedissequamente;